il senatore Tosato richiama l'attenzione del Ministero dell'interno sulla possibile istituzione di una sede di distaccamento permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel Comune di Dolcè, in provincia di Verona, anche in considerazione delle interlocuzioni già avvenute fra le amministrazioni coinvolte. In via preliminare, va segnalato che sono sempre più frequenti le richieste di istituzione di distaccamenti permanenti dei Vigili del fuoco rivolte da vari enti locali al Ministero dell'interno. La maggior parte di tali richieste, pur considerate favorevolmente ai fini operativi, non può essere definita a causa delle oggettive difficoltà di individuare le necessarie aggiuntive risorse umane. Nel caso specifico segnalato dall'interrogante, l'esigenza dell'istituzione di un distaccamento con personale di ruolo dei Vigili del fuoco è stata manifestata diverse volte nel corso del tempo sia dai residenti che dagli amministratori dei Comuni della Valpolicella, nonché da quelli dei Comuni ad essi limitrofi. I sindaci del territorio interessato hanno assicurato l'immediata disponibilità di un immobile sito nella zona industriale di Volargne, frazione del Comune di Dolcè, assicurando altresì l'impegno economico finanziario per gli adeguamenti tecnico-strutturali della potenziale futura sede dei Vigili del fuoco eventualmente necessari. Tale struttura, esaminata con sopralluogo congiunto del Comune e dei Vigili del fuoco stessi, è stata ritenuta idonea per quanto attiene agli spazi, pur necessitando di alcuni lavori di adeguamento. La soluzione prospettata consentirebbe l'apertura immediata del distaccamento fino all'edificazione di una sede definitiva in un'area che le amministrazioni comunali interessate hanno manifestato la volontà di rendere disponibile gratuitamente. Comunico che la richiesta in questione è stata valutata positivamente. Nei prossimi mesi, perciò, sarà possibile procedere alla decretazione del distaccamento, il cui organico sarà potenziato con nove capisquadra nell'anno in corso e completato nell'anno 2024 con ventiquattro Vigili del fuoco. Segnalo anche che, per quanto concerne il personale dei Vigili del fuoco operanti in provincia di Verona, il comando dei Vigili del fuoco di Verona conta, oltre che sulla sede centrale, su quattro sedi distaccate, una delle quali presso l'aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona, l'operatività della quale è limitata all'aeroporto stesso, e le altre nei Comuni di Legnago, Caldiero e Bardolino. Sono presenti inoltre due distaccamenti volontari a Villafranca e a Bovolone.

vorrei su un piano più generale segnalare che l'azione del Governo mira a garantire *standard* qualitativi sempre più elevati nell'attività di soccorso pubblico mediante il potenziamento e la valorizzazione delle risorse umane del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'efficientamento organizzativo e l'ammodernamento delle risorse strumentali. Al riguardo, mi preme evidenziare come, nonostante l'attuale congiuntura economica, con l'ultima legge di bilancio sono state reperite significative risorse finanziarie per le assunzioni delle Forze di polizia e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che hanno consentito l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno in corso, 95 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 e ulteriori somme progressivamente incrementate negli anni, fino a superare i 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2033. Facendo seguito a tale intervento normativo, con decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono state autorizzate assunzioni straordinarie di 1.020 unità di personale nei vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che consentiranno di compensare in parte le carenze che si registrano nel territorio nazionale.

per l'Ovest veronese, ma per tutta la provincia di Verona che - lo ricordo - conta quasi un milione di abitanti. È vero, ci sono quattro presidi, ma giustamente il Sottosegretario ha citato uno di essi situato nell'aeroporto Valerio Catullo e, come tutti sappiamo, quel presidio non può intervenire al di fuori dell'aeroporto, poiché è destinato solo alle emergenze che dovessero verificarsi *in loco*. Quindi, di fatto, i presidi erano tre. Ora assistiamo finalmente a una risposta concreta a una reale necessità del territorio della nostra provincia e a una sinergia perfetta tra amministratori e Governo, perché i quattordici sindaci del territorio coinvolto hanno concordato un'azione comune, si sono confrontati con il Ministero, hanno individuato l'area per realizzare il presidio e l'immobile, al di là delle appartenenze politiche, da parte del Governo c'è stato un intervento molto rapido ed efficace che apprendiamo con favore attraverso la risposta del Sottosegretario. Ricordo che anche recentemente, a febbraio di quest'anno, c'è stato un grave incendio in un'azienda di quel territorio (l'azienda Ci sono stati dei problemi anche nel garantire successivamente la sicurezza dei cittadini in termini sanitari e anche ambientali perché i fumi si sono sviluppati nell'area

Vigili del fuoco del presidio di Verona, quello più vicino, ma naturalmente, se verrà inaugurato un nuovo presidio nella zona della Valpolicella e del Lago di Garda che possa agire su quel territorio, avremo interventi più rapidi che limiteranno i danni, quindi, sottosegretario Molteni, io la ringrazio. Ringrazio il Governo perché siete stati efficaci, concreti e rapidi nel dare una risposta

foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come correttamente osservato dall'interrogante, la presenza invasiva e l'anomala proliferazione della specie aliena granchio blu nei mari antistanti le coste nazionali rappresentano una questione che merita particolare attenzione per i gravi danni prodotti alla molluschicoltura e al relativo comparto. La migrazione di questa specie aliena nel mar Mediterraneo ed in particolare nel mar Adriatico è dovuta prevalentemente all'aumento della temperatura dell'acqua marina a seguito dei cambiamenti climatici, che in presenza di acque calme o poco profonde rappresentano l'*habitat* ideale per la sua riproduzione e crescita. Il granchio blu, che si riproduce in modo incontrollato anche grazie all'assenza di antagonisti marini naturali, è considerato tra le cento specie più invasive del Mediterraneo dell'Adriatico ed ha già interferito con gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche autoctone. Si tratta di una specie predatoria voracissima di pesci, molluschi e crostacei, nonché delle specie allevate dalle imprese di acquacoltura e molluschicoltura. Dallo scorso mese di maggio, subito dopo la prima alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, il granchio blu si è moltiplicato a dismisura nella Sacca di Goro, tra le foci del Po, di Volano e del Po di Goro, in provincia di Ferrara, tra i Comuni di Goro e Comacchio dove viene prodotto circa il 55 per cento delle vongole veraci consumate in Italia, risorsa su cui si fonda l'economia della zona, per un valore di circa 100 milioni di euro. Anche le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Toscana hanno subito l'invasione del granchio blu, che sta impattando non solo sugli allevamenti, ma anche su altre specie ittiche come ad esempio l'anguilla. Considerata la rilevanza della problematica si è reso necessario intervenire con urgenza, consentendo anzitutto il prelievo massivo della risorsa, in un primo momento autorizzando le imbarcazioni a supporto degli impianti di acquacoltura dell'Emilia Romagna con nasse e attrezzi da posta che, anche se non iscritti in licenza, sono nell'ambito della concessione demaniale all'uopo concessa. Successivamente è stata accordata a tutte le imbarcazioni inferiori ai tre GTI iscritte nei compartimenti marittimi dell'Emilia e del Veneto, la possibilità di utilizzare in deroga, entro le 0,3 miglia dalla costa (area dove in genere è assolutamente interdetta la pesca) nasse e reti, anche se non contemplate in licenza. Si calcola che siano state autorizzate almeno 800 barche. Inoltre, per arginare le problematiche connesse alla presenza della specie nei nostri mari, abbiamo immediatamente attivato, a valere sui fondi nazionali, misure di sostegno in favore delle imprese di acquacoltura e della pesca, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta varietà. A valere sul FEAMPA 2021-2027, sono state inoltre attivate ulteriori azioni per il finanziamento di progetti di studio della biologia della specie, finalizzati a controllare l'eccessiva riproduzione del crostaceo e alla creazione di una filiera del granchio blu per il suo utilizzo alimentare (integratori oppure mangimi per acquacultura) e per la commercializzazione e promozione nei confronti del consumatore. Nello specifico, al fine di contenere il fenomeno della diffusione del granchio blu e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, a far data dal 1° agosto 2023, l'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, ha autorizzato la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento della già menzionata specie. Con decreto del Ministro e su segnalazioni delle Regioni sono state individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto. Comunico al riguardo che, in data 27 settembre, il Ministro ha provveduto a caricare nell'apposita piattaforma comunitaria denominata SANI 2 la documentazione relativa al decreto ministeriale citato, che la Commissione dovrà valutare ai fini dell'approvazione del nuovo regime di aiuto. Saranno ammissibili al rimborso i costi sostenuti per gli interventi attuati per la cattura e lo smaltimento del granchio blu. Inoltre, al fine di accelerare e snellire la procedura amministrativa, le istanze di rimborso saranno presentate tramite piattaforma *online*. Peraltro, come già anticipato dal ministro Lollobrigida in occasione di un incontro con le principali associazioni del settore avvenuto lo scorso 26 settembre, al fine di dare continuità agli interventi a supporto del settore ittico è stato previsto un intervento aggiuntivo, come indennizzo alle imprese per l'acquisto di strumenti

ovvero legge di bilancio 2021 e legge pluriennale di bilancio per il triennio 2021-2023, recante criteri e modalità di utilizzazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Informo al riguardo che è in corso di predisposizione un decreto che stanzierà 10 milioni di euro per sostenere una rapida ripresa del settore, indennizzando le imprese per la perdita parziale del prodotto seminato e/o immesso nell'anno 2022 e per l'acquisto di strutture fisse e mobili installate per la protezione degli allevamenti. Inoltre, in data 27 settembre è stato approvato, in sede di conversione del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, un emendamento, nella 9a Commissione del Senato, che prevede l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 500.000 euro, da assegnare alle imprese colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del granchio blu, per un esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti alle suddette imprese, anche per i loro dipendenti. Riguardo all'opportunità di adottare una strategia di più ampio respiro per il contenimento della popolazione del granchio a tutela delle imprese e dell'occupazione, informo l'interrogante che per le problematiche riguardanti la sospensione dei mutui e l'accesso al credito stiamo lavorando per equiparare le regole del mondo agricolo anche a quelle della pesca. Prevediamo un confronto costruttivo con ABI per poter intervenire su questi aspetti. Ciò permetterebbe di semplificare l'accesso ai finanziamenti e di garantire gli stessi diritti degli agricoltori, anche con la possibilità di riconoscere lo stato di calamità. I primi risultati li abbiamo ottenuti nel corso dell'ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell'agricoltura e della pesca, dove abbiamo ottenuto la deroga alla pesca a strascico entro le tre miglia. Questo risultato permetterà di avviare un piano sperimentale di contrasto alla proliferazione del granchio blu, attraverso cui si cercherà di comprendere il ciclo biologico della specie e di valutarne l'impatto sull'ecosistema, per elaborare una strategia che mitighi il rischio di dissesto ambientale. A tal fine, nel mese di giugno ci siamo confrontati anche con degli esperti statunitensi, che conoscono molto bene la tipologia di specie e ne gestiscono da tempo la filiera, recuperando ulteriori considerazioni, in particolare sulle modalità di cattura. Occorre tenere presente che, data la novità del fenomeno, la costruzione di una filiera solida richiede tempo e un'analisi approfondita del mercato. Da qui, la necessità di mantenere un confronto continuo con tutti gli attori interessati. Assicuro infine che il Governo è determinato a sostenere questo settore in una sfida cruciale e continuerà a lavorare in stretta collaborazione con le associazioni per affrontare efficacemente la diffusione del granchio blu e per contrastarne gli effetti.

sicuramente nell'immediato, come lei ha ben sottolineato, servono soldi, servono risorse, servono sostegni concreti e immediati alle imprese ai lavoratori del settore, perché parliamo di migliaia di posti di lavoro. Pertanto, questa è sicuramente un'azione che ci vede assolutamente

sono diventati anche nostri concorrenti e competitori, anche perché hanno abbassato notevolmente il prezzo di questo granchio blu, così violento e aggressivo, che prolifera anche in maniera molto rapida, ma che ma che quando è arrivato nei nostri ristoranti ha incontrato subito la concorrenza sleale da parte di altri Paesi del Mediterraneo, come la Grecia e la Croazia. Con la mia interrogazione ho sottolineato

hanno il timore che, nella prossima estate, già nel 2024 (quindi tra pochi mesi), quando si riaprirà la stagione, potrebbero non avere più quelle risorse alimentari che sono così fondamentali in quel territorio (ma anche le anguille e altri pesci e molluschi importanti) proprio perché hanno svuotato completamente questi mari. Signor Sottosegretario, mi rivolgo a lei, chiedendo anche un'azione strategica di ampio respiro.

un nuovo equilibrio tra predatori, pesci e molluschi che già hanno lì un *habitat* naturale e amico. invece che molte di queste specie sono già sparite, quindi è saltato anche un equilibrio tra il predatore e l'animale che convive in quell'ambiente. Serve almeno il doppio o il triplo di riserve marine. quindi la necessità di ricostruire un *habitat* marino che consenta a quelle zone di ripristinare la natura straordinaria e anche la bellezza romantica e meravigliosa che appartiene a quelle zone lagunari. In conclusione, a mio avviso occorre investire in politiche ambientali concrete, che siano in sinergia con politiche economiche del settore lavorativo e che necessariamente tengano assieme il sostegno economico alle imprese.

Signor Presidente, con riguardo alle misure poste in atto dal Governo per ridurre al minimo i danni provocati dagli incendi boschivi, si premette che il Ministero ha competenza sui piani antincendi boschivi delle aree protette statali, così come previsto dalla legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, mentre gli enti gestori delle aree protette, in attuazione della legge n. 353 del 2000, curano, l'aspetto della previsione e prevenzione. Al fine di coadiuvare gli enti gestori, il Ministero ha redatto uno Schema di piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei parchi nazionali, con relativo manuale di applicazione, e uno Schema di piano AIB omologo destinato alle riserve naturali statali. Per rispondere al possibile aumento degli episodi di incendi boschivi, con il finanziamento del decreto legislativo n. 177 del 2016, il Governo ha previsto l'aumento delle ore di volo sulla linea Erickson S-64F, nonché l'incremento della flotta Canadair CL415 e AB412 destinando circa 14 milioni di euro in totale. Inoltre, per aumentare anche in futuro le ore di volo operative degli elicotteri Erickson, è stato attivato il servizio per l'attività di addestramento degli equipaggi su un simulatore recentemente certificato, che consente di ridurre il numero di voli di addestramento sugli elicotteri ed aumentarne la disponibilità nell'arco della giornata per gli interventi di emergenza. Al fine di garantire una migliore tutela delle aree protette, va anche segnalato il progetto Presidi rurali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volto a garantire una più diffusa presenza del Corpo nelle aree più interne del Paese e una maggiore tempestività negli interventi, con la previsione di nuovi presidi dedicati in via prioritaria, nei periodi di maggior rischio di incendi boschivi, con personale addestrato ed attrezzato in maniera più specifica per questo tipo di attività. L'obiettivo potrà essere raggiunto in diversi *step* che porteranno a regime, con un adeguato aumento di organico, 31 presidi previsti nell'arco di un triennio. Nell'estate del 2023 ne sono stati attivati 19 sul territorio nazionale, all'interno o in prossimità di parchi nazionali e aree protette regionali, in contesti caratterizzati anche da popolamenti forestali di rilevante valore ambientale ed esposti a incendi di interfaccia urbano-rurale. Al riguardo, si rappresenta che il Ministero, oltre a promuovere la collaborazione tra le istituzioni protagoniste nel contrasto al fenomeno degli incendi boschivi partecipando attivamente ai tavoli tecnici nazionali, ha finanziato e finanzia azioni di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi con diversi programmi, tra cui Parchi per il clima, destinato ai parchi nazionali, UNESCO per il clima, destinato ai siti UNESCO, e il Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali, volto al recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi attraverso azioni in linea con la tutela e la conservazione della biodiversità nelle aree protette percorse dal fuoco.

euro. L'incidenza del fenomeno, che abbiamo riportato in modo molto dettagliato in questa interrogazione, è in significativa crescita. Dal 2011 abbiamo registrato il picco massimo degli ultimi quindici anni e nel 2022 la superficie bruciata è stata superiore alla media, a far data dal 2006. una semplice proporzione - come suggerisco al Ministero - tra le risorse che c'erano, quelle che ci sono, la superficie che è coinvolta dagli incendi oggi e quella che era coinvolta poco tempo fa. Tutto questo a far fronte di mezzi dedicati alla Protezione civile, comparto della Difesa, Vigili del fuoco, Arma dei carabinieri e velivoli cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito del progetto "rescEU", assolutamente non sufficienti. Anche a fronte della strutturale carenza di mezzi, le politiche del Governo dovrebbero essere fortemente incentrate sulla prevenzione, con la concentrazione di risorse umane ed economiche in linea con la normativa di settore. Mi consenta da questo punto di vista di dirle anche una cosa che attiene a questa interrogazione e allo specifico del confronto tra Parlamento e Governo, signor Sottosegretario: questa interrogazione, che hanno firmato diversi colleghi, è dello scorso luglio ed era riferita all'estate. Ci confrontiamo oggi, quindi è del tutto evidente che è un confronto postumo,

Da questo punto di vista, l'intenzione preventiva della nostra interrogazione e della nostra sollecitazione appare del tutto vanificata. In particolare, però, in risposta al picco degli incendi boschivi del 2021, il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, ha recato disposizioni per il contrasto agli incendi, promuovendo il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento delle capacità operative.

D'altra parte, parliamo di un fenomeno in crescita e su tutto il territorio nazionale. In particolare, queste risorse ricadevano nei territori della Strategia nazionale delle aree interne (SNAI) e sulle isole minori, anche ad azioni di prevenzione, come il fuoco prescritto, che consiste nell'utilizzo scientifico e pianificato del fuoco durante la stagione invernale da parte di persone qualificate, utile a ridurre l'accumulo della vegetazione infiammabile. Insomma, gli strumenti normativi e finanziari ci sono. Andrebbero potenziati, ma il Governo non può ignorare questo tema, che molto ha a che fare anche con i cambiamenti climatici. Qui è evidente che non aiuta la convinzione o comunque il cedimento all'idea che, tutto sommato, i cambiamenti climatici non ci siano, i loro effetti siano trascurabili o che addirittura siano un pezzo della propaganda, perché è evidente che, se ci si convince che questo fenomeno drammatico e globale non potenzia anche problematiche specifiche, come l'aumento degli incendi boschivi, poi non si ha la stessa determinazione nell'intervenire. La tutela del territorio, i cambiamenti climatici, ma anche - attenzione - la lotta alla criminalità da affrontare: lo dico trovandomi seduto vicino alla senatrice Rando, che è coinvolta rispetto a questi fenomeni. Insomma, speriamo che questo tema possa avere in futuro il rilievo che merita nell'agenda di Governo, a differenza di quanto abbiamo sentito oggi in risposta alla nostra interrogazione. Magari mi premurerò, Presidente,

Signor Presidente, gentili senatori, il ritiro sociale, noto con il termine *hikikomori*, appare oggi come un fenomeno in aumento, con un esordio sempre più precoce che comporta un'interruzione del percorso evolutivo e un importante rischio per lo sviluppo degli adolescenti. Il contesto pandemico e il conseguente confinamento hanno gravato in modo specifico su quei ragazzi e adolescenti che già si trovavano in situazioni di isolamento, di autoreclusione in casa o che si erano volontariamente allontanati dai contesti sociali e abituali, inclusa la scuola e i gruppi di pari. A fronte di questo quadro, è necessario mettere in atto azioni di prevenzione e di intercettazione precoce delle situazioni di potenziale fragilità e ritiro sociale, seguite da interventi tempestivi a vario livello, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni, i servizi e i soggetti implicati nel sostegno alla crescita dei bambini adolescenti, riguardando peraltro la competenza di più Ministeri. Infatti, con riferimento alle iniziative di competenza del Ministero della salute, segnalo che quest'ultimo agisce su più fronti, sia con risorse dedicate a interventi di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto al ritiro sociale, sia attraverso protocolli interistituzionali con il mondo della scuola, per la promozione di una cultura e di un'azione conseguente di prevenzione e cooperazione tra tutte le istituzioni, i professionisti e gli adulti di riferimento che si occupano e si prendono cura di adolescenti e preadolescenti, al fine di tracciare buone prassi che accompagnino i giovani nel loro percorso di crescita. Nell'ambito delle attività istituzionali, ad esempio, con l'obiettivo di coordinare e di garantire l'integrazione degli interventi per la tutela e la promozione della salute e del benessere psicofisico, è stato stipulato il protocollo d'intesa a tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione, con validità triennale. Inoltre, nel quadro delle alleanze e sinergie intersettoriali, richiamo il Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, adottato dal Ministero della salute, che individua nella scuola l'ambiente più adatto per riconoscere precocemente i problemi psicologici e comportamentali di bambini e adolescenti, favorendo la possibilità di intervenire tempestivamente. D'altro canto, rappresento che anche il Ministero dell'istruzione e del merito, per quanto di competenza, è impegnato da anni nell'approfondimento delle strategie di prevenzione e contrasto di tali fenomeni all'interno della comunità scolastica, proprio al fine di intercettare e arginare comportamenti a rischio, determinati in molti casi da condizioni di disagio sociale non riconducibili solo al contesto scolastico. Al riguardo, tra le iniziative promosse, segnalo in particolare il progetto "Generazioni Connesse", cofinanziato dalla Commissione europea, quale centro nazionale per la promozione di un uso sicuro e positivo della Rete rivolto a studenti, insegnanti, genitori, enti, associazioni e aziende. la linea di ascolto che, nell'ambito del progetto "Generazioni Connesse", supporta ragazzi e adulti che devono affrontare situazioni difficoltà o pericolo in Rete, garantendo uno spazio di confronto con il personale specializzato. le attività e le campagne di sensibilizzazione e informazione legate ai possibili rischi emergenti nella navigazione in Rete, attraverso le quali si è intervenuti per promuovere la conoscenza tra insegnanti, studenti e genitori del fenomeno del ritiro sociale, come di altri fenomeni derivanti da un uso distorto dello strumento digitale. In ultimo, condivido con l'onorevole interrogante che condizioni di disagio e di malessere dei ragazzi possono essere una delle cause dell'insuccesso formativo e della dispersione scolastica. Affrontare un fenomeno così complesso richiede un approccio multi-fattoriale, in un'ottica di sistema che il Piano nazionale di ripresa e residenza affronta con interventi mirati. Mi riferisco non solo all'Investimento 1.4, finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica, ma anche alla riforma dell'orientamento, che ha portato all'adozione di specifiche linee guida che introducono, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, moduli curriculari di orientamento formativo degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Con le medesime linee guida sono state istituite due nuove figure professionali: il docente *tutor* e il docente orientatore, alle quali il Governo ha dedicato misure di valorizzazione sia economica (con uno stanziamento di 150 milioni di euro previsto dalla scorsa legge di bilancio e ripartito con il decreto ministeriale

A conferma della particolare attenzione che il Ministero dedica alle tematiche richiamate nel presente atto, aggiungo in ultimo che, per contrastare il disagio giovanile e la povertà educativa, con il decreto-legge 123 del 2023 abbiamo introdotto misure volte a rafforzare in maniera complementare e sinergica le azioni previste dal Piano Agenda Sud, che mira a ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali negli apprendimenti nelle Regioni del Mezzogiorno.

inizialmente indirizzata alla Commissione. Quindi grazie per l'attenzione rivolta a un fenomeno che, molto probabilmente, è poco conosciuto nella sua specificità. Nella Nella sua risposta il Sottosegretario ha parlato di disagio giovanile dove c'è una interdipendenza, ma questo è un fenomeno un po' particolare e specifico. Parliamo - come diceva il Sottosegretario nella sua risposta - di ritirati ed eremiti sociali. Nella ricerca che io ho indicato nell'interrogazione si parla di 54.000 adolescenti e si cerca di capire quali sono le cause

ignorata. La stima dell'isolamento volontario nella popolazione adolescente sta sempre di più aumentando. I sintomi - da quello che dicono le ricerche,

in materia di tutela del paesaggio e di conservazione delle antichità e delle opere artistiche e dei beni culturali, nei limiti tracciati dalla Costituzione. Questo Ministero ha un potere di vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), fondazione che ha tra gli scopi istituzionali l'organizzazione delle rappresentazioni classiche presso il teatro di Siracusa; al contrario non svolge la funzione di tutela nel territorio siciliano e quindi sui beni che sono utilizzati dalla stessa fondazione. Non di meno, corre l'obbligo di evidenziare che l'assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana riferisce che non risultano criticità sul monumento e la stessa soprintendenza, con nota del 13 marzo 2023, afferma che non emergono problemi alla *cavea* del teatro prodotti dal carico antropico della stagione appena terminata, né a seguito dell'attività di smontaggio. Per questo motivo è stato autorizzato il progetto di attrezzamento per la stagione estiva 2023, per quanto di competenza della suddetta autorità, sotto il profilo della tutela archeologica e paesaggistica, ai sensi dell'articolo 21 del codice dei beni culturali. Già da anni, per i cicli di rappresentazione del dramma antico e degli altri spettacoli, il teatro viene rivestito da una sovrastruttura in legno che poggia su cuscini di sabbia, con lo scopo di preservarla dall'erosione portata dall'uso e dalla pressione antropica. Dato l'intensificarsi della programmazione artistica e il moltiplicarsi degli eventi portati in scena e, in generale, per il controllo dello stato di salute del teatro, riferisce ancora la soprintendenza che a partire da gennaio 2023 è in corso una campagna di indagini, con l'utilizzo delle più moderne tecnologie e dei migliori professionisti del settore, anche al fine di valutare la compatibilità del suo utilizzo con le attuali condizioni statiche e di conservazione. L'obiettivo è di procedere a un completo intervento di restauro. Risultano inoltre al vaglio del governo regionale soluzioni alternative per contemperare le esigenze di tutela con quelle della valorizzazione e della fruizione del sito archeologico, quali lo spostamento di concerti ed eventi nell'ara di Ierone, all'interno dello stesso parco. Al riguardo è in corso di valutazione la realizzazione di una struttura mobile capace di ospitare circa 5.000 persone.

un teatro scavato nella roccia, a differenza di altri, quindi soggetto, anche per la particolarità della roccia, a forme incisive di erosione, anche di tipo metereologico, e la

Il tema che si è posto, però, è proprio quello di provare, fatte salve ovviamente le competenze regionali, a individuare in qualche modo un trattamento unitario, non solo nella specificità di quella zona, ma in generale, nella fruizione di beni archeologici archeologici che hanno un valore immenso. Ciò significa immaginare una politica di fruizione che sia il risultato di studi sul livello di erosione, di sostenibilità, di tollerabilità rispetto a tutta una serie di fenomeni. È

sono un insieme di articoli che individuano innanzitutto quale debba essere il criterio della valorizzazione e della compatibilità. L'articolo 5 introduce un principio di sussidiarietà, ma anche di sostituzione, laddove prevede che il Ministero eserciti la potestà di indirizzo e vigilanza - come il Sottosegretario giustamente ha evidenziato - ma anche il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. Avrei quindi voluto sapere - e per questo sono parzialmente insoddisfatto della sua risposta quali concrete misure di vigilanza, una volta annunciate queste misure, il Ministero intende realizzare. Secondo me, la vigilanza deve essere di due tipi: ovviamente quella fattuale su cosa si sta facendo e perché, ma anche quella di tipo tecnologico e scientifico, quali strumenti si stanno utilizzando per la misurazione, in quanti percorsi possibili anche di monitoraggio e quali sono le risposte migliori che si possono dare. si pone un tema di tutela dei beni culturali, di tutela del turismo, ma anche di individuazione di nuove aree - come è stato detto - e anche di strumenti legislativi che possono contemperare le due esigenze, come chiedevamo nella nostra interrogazione.

la cultura*. A seguito della caduta di calcinacci di una parte del sottotetto del porticato esterno dell'Archivio centrale di Stato, si chiede di conoscere l'intenzione del Governo al fine di assicurare condizioni di sicurezza e dignitose per lavoratori, studiosi, appassionati, ricercatori e cittadini che intendono esercitare il proprio diritto di accedere e fruire dell'immenso patrimonio culturale espresso dalla documentazione conservata all'Archivio centrale. In via preliminare, sulla caduta nel mese di maggio scorso di una parte del sottotetto del porticato esterno è necessario precisare che l'immobile è di proprietà dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL), e da questi dato in locazione all'Archivio centrale dello Stato. Pertanto, la responsabilità contrattuale della manutenzione straordinaria ricade principalmente sull'Istituto previdenziale. Per questa ragione, l'Archivio ha sempre segnalato qualsiasi problematica muraria o di altro genere all'ente proprietario, cui è stato fornito riscontro con lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare dell'edificio centrale e laterale. L'INAIL ha già avviato un progetto di riqualificazione di tutto l'immobile, che riguarderà la parte muraria esterna identificata come lotto 1, il cui bando di gara è già stato pubblicato, nonché di tutti gli impianti della struttura identificata come lotto 2, quest'ultimo in fase di progettazione esecutiva. Sul presunto malfunzionamento da diversi mesi dell'impianto di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria, si tiene a precisare che non risulta che alcun dipendente o utente abbia patito il freddo durante l'inverno. alle segnalazioni ricevute dall'ufficio tecnico dell'Istituto, le stesse sono state prontamente prese in carico e risolte in breve termine. Il sistema di riscaldamento, in particolare, ha funzionato per tutto il periodo invernale e solo agli inizi del mese di febbraio sono state riscontrate alcune anomalie riguardanti la natura tecnica dell'impianto sotto manutenzione della ditta affidataria del servizio. Tali circostanze, comprese ulteriori problematiche tra cui diverse infiltrazioni di acqua, sono state segnalate all'INAIL, a cui sono seguiti il riscontro e il sopralluogo del 30 marzo 2023. A fronte del citato sopralluogo con i responsabili INAIL, sono seguiti lettera di segnalazione e interventi vari sull'edificio dell'Archivio centrale dello Stato, comprensiva della problematica riguardante la caldaia. In particolare, in un'ottica di programmazione e sicurezza del sistema di riscaldamento, si è provveduto a verificare le condizioni delle caldaie che alimentano l'impianto di riscaldamento. Dal sopralluogo è emerso che, delle tre caldaie presenti, due non sono funzionanti e una terza è più volte messa in blocco causando la continua interruzione del regolare flusso di riscaldamento dell'intero immobile. Inoltre, le stesse caldaie e il locale tecnico non presentano sistemi di sicurezza adeguati. La ditta di manutenzione ha precisato il suo malfunzionamento specificando l'esigenza di un intervento straordinario prima di una nuova eventuale accensione. Sullo stato attuale dei termosifoni presenti al piano secondo dell'edificio centrale, è stata segnalata la presenza di numerosi termosifoni, così come verificato in presenza, il cui stato è ormai obsoleto e molti dei quali presentano copiose perdite di acqua, a cui si è dovuto provvedere con la chiusura degli stessi. Altri invece presentano precarie condizioni in cui è evidente la presenza di ruggine e sono prossimi a ulteriori perdite. Sono stati chiesti tempestivi interventi per garantire il corretto funzionamento dell'impianto prima della stagione invernale, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dell'attività dell'Archivio centrale. A fronte di tale segnalazione, l'INAIL ha dato riscontro con lettera del 3 maggio 2023, dove è stato rilevato che nel corso del sopralluogo si è inoltre accertata la necessità di sostituire una delle due pompe dell'impianto di riscaldamento. L'intervento è già stato programmato in fase di affidamento. L'esecuzione delle opere è prevista in data antecedente alla prossima stagione. Pertanto, per quanto concerne il riscaldamento, l'Istituto ha garantito il funzionamento durante l'inverno effettuando tutte le dovute segnalazioni di competenza e ha programmato l'intervento prima dell'inizio della nuova stagione invernale. Per quanto concerne l'impianto di raffreddamento, nonostante le numerose difficoltà tempestivamente segnalate all'INAIL, l'impianto di raffreddamento attualmente è in funzione. In ogni caso, a causa delle diverse problematiche rilevate, l'Istituto non ha mai interrotto il servizio all'utenza, garantendo l'apertura per le intere giornate settimanali e sempre in condizioni di piena sicurezza. Signor Sottosegretario, la ringrazio per la risposta e le dico la verità: mi dovrei dichiarare assolutamente se questa fosse un'assemblea di condominio, perché la sua disamina è stata analitica, precisa, perfetta, anche con un livello di dettaglio devo dire - di piena soddisfazione. Ma - ahimè - non stiamo parlando in una assemblea di condominio: siamo nell'Aula del Senato e stiamo discutendo non soltanto di questioni meramente immobiliari - caldaie, radiatori, condizionatori, che per carità sono importantissimi

anche fisicamente oltre che simbolicamente, rappresenta un po' la nostra memoria, il luogo nel quale noi raccogliamo tutte le tracce di ciò che siamo stati e dunque di ciò e probabilmente anche di ciò che saremo. È evidente che su quella memoria abbiamo costruito la nostra storia, costruiamo la nostra identità nazionale e in un certo senso anche il nostro futuro. Abbiamo bisogno che quell'Archivio centrale dello Stato non sia non sia considerato soltanto un immobile che dobbiamo manutenere, come manuteniamo un negozio o un appartamento: è un luogo che ha - mi perdoni se utilizzo una parola forse importante - una solennità che è ai limiti della sacralità.

dobbiamo mettere nelle condizioni non soltanto chi vi lavora - ovviamente come in tutti i luoghi di lavoro e in questo in particolare - ma anche chi in esso studia e chi vuole fruire di quella memoria

che consentano una ricerca per esempio storiografica di altissimo livello; che tutta l'infrastruttura sia costruita in modo da far sì che chi lavora su quella memoria possa farlo nella condizione di massima efficienza ed efficacia. Vorrei insomma che

anche ispirate a un senso di visione strategica che io, Sottosegretario, nella sua risposta francamente non ho colto. Sappiamo bene che la nostra Costituzione promuove la cultura e la conoscenza e direi che mai come in questo tempo così veloce e così liquido la memoria rappresenta un'ancora rispetto ai valori che quella Costituzione incarna: la nostra democrazia, le nostre libertà, i nostri diritti se vuole - mi perdoni se da una questione immobiliare faccio un salto così alto - la nostra collocazione internazionale e i valori europei. Tutto questo sta dentro quell'immobile. Quindi, sentire che sono caduti calcinacci o che la temperatura dell'ambiente non è quella giusta, ci costringe a degradare un discorso che dovrebbe essere

signor Sottosegretario, io non sono soddisfatto e utilizzo questa occasione per spronare davvero il Ministero della cultura e il Governo a prendersi cura di questo gioiello, di questo luogo così prezioso e di custodirlo con la cura che è necessaria e che - mi perdoni - dalle sue parole oggi non ho colto.

Innanzitutto, si fa presente che l'Archivio di Stato di Roma ha occupato la sede di via Galla Placidia in regime extracontrattuale, con un canone di circa 700.000 euro annui, e che la rinegoziazione di tale canone al prezzo stabilito dall'Agenzia del Demanio ha inizialmente incontrato il rifiuto risalente all'aprile 2021 della proprietà. Si fa presente, altresì, che l'Archivio di Stato di Roma è destinatario in uso governativo di una nuova sede, sita in via dei Papareschi, di circa 13.000 metri quadrati, assegnata dal Demanio nell'anno 2020 per lavori di adeguamento strutturale, al termine dei quali tale sede ospiterà la documentazione attualmente conservata a via Galla Placidia. Nelle more della conclusione dei lavori e della mancata rinegoziazione del canone di locazione, il Ministero ha sospeso l'utilizzo delle risorse finanziarie, pari a 466.896 euro, destinate all'adeguamento antincendio della sede di via Galla Placidia, non ritenendo opportuno intervenire su un edificio in occupazione extracontrattuale. A sua volta, il direttore dell'Archivio di Stato di Roma, essendo anche datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha ritenuto di dover chiudere la citata sede, sia agli utenti esterni che al personale dell'Archivio, per garantire agli stessi le necessarie misure di sicurezza. Dopo un incontro con le organizzazioni sindacali per esporre le motivazioni della chiusura e trovare soluzioni che garantissero la continuazione della consultabilità dei documenti, la Direzione archivi ha provveduto a contattare direttamente sia la proprietà che l'Agenzia del Demanio competente, al fine di addivenire a una soluzione e dunque evitare lo spostamento della documentazione, dato che, nel frattempo, la proprietà di via Galla Placidia, a dicembre 2021, aveva rettificato la sua posizione di diniego al rinnovo del contratto di locazione al prezzo stabilito dal Demanio, che era appunto di euro 446.352 euro, e si è resa disponibile a rinegoziare il canone stabilito. Grazie all'impegno del Ministero, la situazione di extracontrattualità dei locali archivisti è cessata, in quanto il 31 agosto 2023 è stato finalmente rinnovato, per nove anni, il contratto di locazione, per un importo complessivo di euro 446.352 più Iva, con la Società Generale Costruzioni Ricostruzioni, So.Ge.Co.Ri., proprietaria dell'immobile, quella che inizialmente non aveva accettato la rinegoziazione del canone. Il 18 settembre 2023 il contratto di locazione è stato trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Il 26 settembre il Ministero ha comunicato al segretariato regionale del Ministero della cultura del Lazio di riprendere le attività necessarie per l'adeguamento antincendio della sede succursale dell'Archivio di Stato di Roma di via di Galla Placidia. Sulla base della richiesta dell'Archivio di Stato di Roma, la Direzione generale competente ha altresì messo a disposizione le risorse per l'affidamento del servizio navetta per la presa e ricollocazione del materiale per la consultazione da via Galla Placidia ai locali di via del Senato, sede principale dell'Archivio di Stato di Roma. Non appena saranno risolte le problematiche legate all'impianto antincendio, si potrà finalmente riaprire la sede, che nel mentre resta temporaneamente chiusa a garanzia e a tutela di utenti e lavoratori.

C'è un tema enorme che riguarda la riapertura di quella sede in condizioni di sicurezza per gli studiosi che vi lavorano e per l'utenza che vi può accedere. C'è un grandissimo patrimonio e - prima ne abbiamo parlato l'Archivio di Stato si tratta di infrastrutture della conoscenza essenziali alla ricerca, ma anche ai tecnici, cioè alla contemporaneità. Il patrimonio dell'Archivio di Roma di via Galla Placidia riguarda lo lo Stato postunitario, lo Stato Pontificio: è davvero un *unicum.* Rimane il fatto che per questi mesi, non si sa fino a quando, la sede sarà chiusa. sarà chiusa. È vero che dal 9 ottobre sarà riattivata la possibilità di accedere alla documentazione dell'Archivio, ma noi dobbiamo assicurarci che al più presto possa essere riaperta quella sede, anche perché l'edificio di via dei Papareschi avrà bisogno di molti anni anni di lavori per poter essere aperto al pubblico. Mi dichiaro quindi parzialmente soddisfatta perché c'è stato bisogno di questo allarme. Mi fa piacere sentire

a un fatto accaduto ieri durante una ricostruzione abbastanza curiosa del mio operare nelle Commissioni riunite 9a e 10a, quando sono stato accusato di aver leso di fatto le prerogative parlamentari di un'esponente del MoVimento 5 Stelle.

nessuno, o meglio la collega che si lamenta non ha visto nulla e anzi cita un labiale, mentre in momenti concitati di solito dovrebbe essere l'audio quello che colpisce di più, e non il labiale. Tuttavia, giacché non c'è alcuna menzione, perché non c'è nulla nemmeno nei verbali, quello che mi preme sottolineare non è tanto il commento a queste ricostruzioni, quanto il fatto che io non sono uso - e credo che ciò sia assolutamente testimoniato anche dagli atti, non dal sentito dire o dalla mia autoreferenzialità - ledere alcuna prerogativa parlamentare. Lo raccontano gli atti; lo racconta proprio ieri un provvedimento, quello sulle materie prime rare, sul quale, grazie al tanto lavoro di maggioranza e opposizione, siamo riusciti ad avere un testo unificato che è espressione delle volontà e dei *desiderata* di tutti i Gruppi. Pertanto, nella stessa giornata nella quale io avrei pregiudicato le

anche in Aula mi si ringrazia per il mio operato e il grande lavoro; non ultimo il provvedimento sugli incentivi alle imprese della settimana scorsa, nel quale

alle quali risponderanno il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso. La senatrice Naturale

del fungo della peronospora. Tale congiuntura deriva sicuramente dai cambiamenti climatici, perché mai a memoria dei nostri genitori si era affrontata una situazione del genere. La peronospora è una fitopatia propria della vite, quindi è impensabile che gli agricoltori non abbiano messo in atto

perché purtroppo questi danni non sono un fatto occasionale, non si può parlare di crisi di impresa, ma bisogna trovare delle soluzioni pregnanti e strutturali. Anche la Banca centrale europea non aiuta, con i tassi sui mutui che sono assolutamente proibitivi e che mettono in ginocchio i produttori anche nell'affrontare i futuri costi per la gestione e di una futura campagna viticola. Pertanto, chiedo anche che si possano sbloccare i fondi di riserva di crisi, ad esempio, per dare un sostegno utile a fondo perduto, con la sospensione di mutui. Il settore vitivinicolo

Devo dire che le constatazioni che lei ha fatto sono corrette: quest'anno ci troviamo di fronte ad un'aggressione della peronospora come non si registrava da tempo e a una riduzione della produzione che l'osservatorio vendemmiale Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini stima

7 milioni di intervento che sono solo un inizio e che spero il Parlamento, già durante la legge di stabilità, potrà implementare. Noi proveremo a farlo, nell'ambito delle risorse disponibili, anche nella fase di redazione del provvedimento, ma bisogna tener conto che non sempre - questo è un dato oggettivo che dobbiamo valutare - la riduzione della produzione corrisponde a una riduzione del valore. Evidentemente noi dobbiamo intervenire per ripagare le imprese della perdita di valore più che della perdita di produzione, anche in considerazione del fatto che c'era un problema interconnesso al sistema vino che lei, senatrice, ben conosce, che è lo stoccaggio di un quantitativo di vino eccessivo prodotto lo scorso anno. È per questo che nel decreto-legge abbiamo voluto prevedere anche un intervento normativo, mi sembra a firma del collega De

le perdite per le aziende e mantenere sul mercato una quantità di vino italiano importante. Dobbiamo aspettare l'imbottigliamento e la vendita per capire la perdita di valore, sulla quale immagino insieme avremo più occasioni di intervenire. Certamente teniamo conto anche del fattore che lei richiamava delle imprese biologiche e anche nel decreto che il Ministero provvederà a discutere con la Conferenza delle Regioni e con le associazioni di settore valuteremo la tipicità e la tipologia delle diverse imprese e anche la possibilità di intervenire nella fase preventiva per cercare di limitare i danni utilizzando le buone pratiche che la PAC prevede e che purtroppo sono limitate per le aziende biologiche al solo utilizzo del rame. Abbiamo provato a chiedere la deroga alla Commissione europea, che però ci ha dato parere negativo e di questo non possiamo che tenere conto. possiamo che tenere conto. Questo Parlamento è stato avanguardia in Europa nella discussione sulla difesa, al netto di pesticidi, delle nostre colture, attraverso le tecnologie evolutive avanzate, che nulla c'entrano con gli OGM, ma che invece accelerano alcuni processi di rafforzamento delle colture, proteggendo le piante dalle vecchie e nuove aggressioni, dalle fitopatie, dal cambio climatico e da quanto noi vorremmo evitare di curare con gli agrofarmaci, che però talvolta sono l'unica soluzione attuale. Abbiamo lavorato sugli OCM del vino, che evidentemente tengono conto in maniera preferenziale del biologico, perché riteniamo che tutte le produzioni che salvaguardano la qualità, senza dover utilizzare agenti esterni, siano da prediligere e preferire rispetto ad altro. Abbiamo anche cercato - per dirla in maniera un po' cruda - di svuotare i cassetti del Ministero, come anche lei nel suo quesito ci invita a fare, per trovare risorse interne. Siamo riusciti ad intervenire con 100 milioni immediatamente in sostegno della Regione Emilia-Romagna, con un fondo alluvionale e con fondi propri del Ministero, così come abbiamo trovato 13 milioni per affrontare la questione emergenziale del granchio blu che aggredisce le aziende di pesca italiane, in particolare dell'acquacoltura, così come abbiamo ritrovato nei fondi interni del Ministero 7 milioni per la peronospora (per ora). Questo è quello che abbiamo fatto con fondi che abbiamo utilizzato, ma che non era previsto venissero usati per cose che non potevamo conoscere, proprio perché il cambio climatico da un lato e una serie di altri fattori stanno facendo nascere una serie di emergenze. Chiudo con un invito invito ad affrontare questo tema con la valorizzazione di un *asset* strategico, come quello delle produzioni vinicole, che sono e continuano ad essere il gioiello della nostra produzione italiana: è per questo che in ogni campo crediamo ancora oggi opportuno tentare di proteggerle e valorizzarle.

Non gli arriverà dunque nulla, in definitiva, perché questi sono 7 milioni di euro da spalmare in tutta Italia. Anche sul biologico speravo in una risposta che fosse di maggiore pregnanza rispetto a questo settore, in vista della tutela dei dei prodotti di nicchia e della tutela anche della biodiversità e dell'ambiente, in quelle che sono produzioni sostenibili che devono entrare di forza e di prepotenza nel piano vitivinicolo. L'impegno del Governo dovrebbe essere strutturale nel garantire un futuro alle aziende e dovrebbe essere

signor Ministro, la produzione di carne bovina in Italia corrisponde al 50 per cento del fabbisogno. Il grado di produzione interna sale poi al 74 per cento se consideriamo anche i capi importati e ingrassati fino a sei mesi in allevamenti. In ogni caso, il 26 per cento della carne alimentare che abbiamo nel nostro Paese è importata come carne macellata. Negli allevamenti italiani sono ormai delle eccellenze le razze autoctone, iscritte nei libri genealogici. Tra queste ricordiamo: la razza piemontese, la chianina, la marchigiana, la maremmana, la romagnola e la podolica. Le razze da carne autoctone iscritte nei libri genealogici contano oltre 530.000 capi allevati qui in Italia, di cui 268.000 sono vacche; sappiamo bene che, oggi come oggi, le vacche sono per il 98 per cento vacche nutrici. Questi allevamenti contribuiscono all'8 per cento del fabbisogno di carne bovina nazionale. Il tema è che il mercato delle razze bovine autoctone da carne è in crisi. Il crollo dei prezzi di vendita sta mettendo a serio rischio di sopravvivenza gli allevamenti italiani, che rappresentano l'anello più debole della filiera. In particolare, la razza bovina piemontese, che è una tra le razze da carne autoctone più diffuse nel nostro Paese, conta circa 340.000 capi; 4.150 sono gli allevamenti, il 60 per cento dei quali è presente in Provincia di Cuneo, per un giro d'affari che supera il miliardo di euro. Nella nostra Provincia piemontese, poi, si è sviluppata un'importante attività di alpeggio, la cosiddetta transumanza, dove lavorano 1.300 famiglie con 2.600 addetti, tra cui anche molti giovani. Nella stessa Provincia di Cuneo è presente l'Associazione nazionale bovini razza piemontese, che è vigilata dal Ministero e anche in parte finanziata. In mancanza di un'adeguata valorizzazione, la razza piemontese rischia di essere compromessa tra le eccellenze agroalimentari italiane, creando le condizioni per aumentare le importazioni di prodotti dall'estero. Lei sa bene che, negli ultimi anni, l'aumento dei prezzi di produzione è stato di oltre il 50 per cento, a fronte del prezzo dell'animale alla stalla

Occorre anche ricordare la valenza dei libri genealogici, gli ispettori e la capacità di mantenere le razze all'interno di certi crismi e soprattutto di certe garanzie. Noi siamo a chiederle, signor Ministro, se il Governo voglia mettere prontamente in atto tutti gli interventi necessari al sostegno di tutte razze da carne autoctone italiane, ma soprattutto di quella piemontese, che ha una sua importanza particolare, prevedendo anche l'istituzione di un apposito fondo (siamo in vista della legge di bilancio). Qualcosa è già stato fatto in passato, però chiediamo a lei di dare una risposta a tutti questi allevatori impegnati.

io in apertura sottolineo come auspicio tenda a proteggere produzioni di eccellenza, come una delle migliori carni prodotte da una razza come quella piemontese, nell'ambito di una ricca offerta genetica italiana, che però nel quadro che lei ricordava certamente vede eccellere la Fassona di razza piemontese che evidentemente è considerata tra le più prestigiose. della sovranità alimentare e delle foreste, abbiamo sostenuto il riconoscimento delle IGP e il sistema della qualità nazionale di zootecnia. Tali decisioni rientrano nel più ampio impegno del Governo diretto a contrastare gli allevamenti intensivi, creando le condizioni affinché l'attività zootecnica possa avvenire nel rispetto del benessere animale per tante ragioni; per l'animale stesso, ma anche per la qualità dei prodotti. Qualche giorno fa, a Bra, abbiamo ascoltato un intervento importante, sul quale anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, si è impegnato a tutelare e sviluppare i prati stabili; un'iniziativa interessante che garantisce la possibilità di avere un equilibrio ambientale e produzioni di grande qualità. Lei ricordava la transumanza, un altro elemento tipico e tradizionale, ma di allevamento corretto nel rispetto della vita dell'animale. Certo, gli animali in quella fase vanno protetti anche dai grandi carnivori e dalle aggressioni che possono rilevarsi a danno di quell'allevamento tradizionale che deve e può rafforzare la filiera, con quel valore aggiunto dato proprio dalla qualità delle nostre produzioni. altri elementi che lei ha citato correttamente, voglio ricordare che abbiamo stanziato con decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, risorse per 3 milioni di euro nel 2023 e 5 milioni nel 2024, finalizzate a sviluppare l'operatività della banca dati unica zootecnica, strumento imprescindibile per la mappatura chiara del patrimonio zootecnico nazionale, che serve evidentemente allo studio e al rafforzamento delle razze. Siamo consapevoli che l'attività di miglioramento genetico rappresenta un investimento strategico di lungo periodo, con effetti lungo tutta la filiera produttiva. Per questa ragione il Ministero eroga contributi alle associazioni nazionali di allevatori riconosciuti quali enti selezionatori. Negli ultimi anni, fino al 2024, il sostegno all'attività dei programmi genetici è stato attuato anche con il programma di sviluppo rurale 2014-2022, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e la biodiversità animale attraverso un sistema innovativo integrato di assistenza zootecnica. Le associazioni degli allevatori sono dunque beneficiarie di finanziamenti, come da lei ricordato, che consentiranno di ultimare lo sforzo e la caratterizzazione delle razze presenti sul territorio nazionale nonché di proseguire le attività di assistenza agli allevatori per quanto relativamente agli accoppiamenti programmati, al fine di valorizzare al meglio il potenziale genetico degli animali allevati e migliorare le *performance* riproduttive. L'obiettivo è quello di riorganizzare il sistema di allevamento puntando sulle specializzazioni.

incentivare ed implementare non solo la produzione finale, ma anche l'allevamento e la crescita di filiere che siano idonee a garantirlo. Questi obiettivi che ci siamo posti, che fanno parte, evidentemente, di una cultura che ritiene l'allevamento, la pesca e l'agricoltura centrali nel nostro sistema di sovranità alimentare, per garantire una produzione che prescinda da eventi contingenti, come le pandemie e le guerre, che purtroppo sono tornate alle nostre porte, vedono nell'allevamento delle carni rosse e anche delle mucche da latte un imprescindibile investimento, che spero verrà implementato, come lei ricordava, da azioni sinergiche tra Governo e Parlamento, per poter avere le risorse necessarie per migliorare ancor di più questo impegno, che ho provato, per grandi linee, a descrivere e che, ovviamente, prevede tra le misure l'investimento strategico e importantissimo della PAC 2023-2027, con 37,2 milioni di euro annui di stanziamento a tutela e a difesa del nostro sistema di allevamento.

che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti, bevande e mangimi sintetici. Questo è stato un passaggio fondamentale, ma insieme crediamo che a ciò vada collegato direttamente il sostegno alle filiere produttive. Qui vengo a parlare del tema delle razze autoctone. Come lei ha spiegato bene in precedenza,

perché soffrono in un momento di grandissima difficoltà. Credo che gli allevatori italiani possano contare su di lei, signor Ministro, sulla sua grande disponibilità, sull'attività della nostra Commissione e su questo Parlamento, perché le risposte che dobbiamo dare a questi allevatori sono importanti, per sostenere il grande sacrificio che fanno ogni giorno. *(Applausi)*.

Presidente, signor Ministro, qualche giorno fa, il 2 ottobre, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha pubblicato una sentenza, come lei sa bene, nella quale chiarisce come il salario minimo fissato dalla contrattazione collettiva non sia esente da una verifica del giudice sulla congruità rispetto ai parametri costituzionali della giusta retribuzione, sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. Nel dettaglio, dopo che il giudice di primo grado aveva dato ragione al dipendente di una cooperativa adibito a mansioni di vigilante in un supermercato di Torino, che lamentava la non conformità all'articolo 36 della Costituzione del suo contratto collettivo nazionale, la Corte d'appello si era in un primo momento fermata, riconoscendo un primato alla contrattazione collettiva. Poi però la Corte di cassazione ha ribaltato la sentenza di secondo grado

del giusto livello di salario, come appunto viene scritto. Quindi, nonostante la libertà negoziale, i contratti collettivi non possono prevedere minimi salariali che non siano proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro e sufficienti ad assicurare «a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa», proprio come prevede il citato articolo della Costituzione. È invece necessario - sottolinea la Cassazione - fissare una cifra che risulti adeguata a queste necessità di base, quindi un salario minimo costituzionale in grado di garantire una vita libera e dignitosa, e non solo non povera. Ministro, evidentemente è proprio a quei contratti che condannano lavoratrici e lavoratori di questo Paese alla povertà. Nonostante il lavoro, sappiamo dai numeri che parliamo di circa 4 milioni di lavoratori al di sotto della soglia

come purtroppo è già accaduto troppe volte nel corso di questi ultimi anni, che il Parlamento arrivi eccessivamente in ritardo su questioni rispetto alle quali invece dovrebbe ribadire tutta la propria centralità e non delegare a nessun altro.

che mi permette di fornire dei chiarimenti in merito all'adeguatezza dei livelli salariali. Preliminarmente, credo sia doveroso per me sottolineare che il disegno di legge citato nell'interrogazione è una proposta di natura parlamentare, il cui *iter* è rimesso, come previsto dall'ordinamento, alla volontà sovrana del Parlamento. Quindi, con riferimento alla richiesta di intervento sulla calendarizzazione del disegno di legge, in qualità di Ministro della Repubblica rappresentante dell'Esecutivo, e per il rispetto che avverto nei confronti delle Assemblee, non ritengo opportuno esercitare alcuna azione in relazione ad atti che sono propri del procedimento parlamentare. In ogni caso, credo che il tema dell'adeguatezza dei livelli salariali sia centrale per la tutela delle condizioni di lavoro e rappresenti una tematica di di grande rilevanza per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla quale certamente pongo la massima attenzione. Per questo motivo credo che il Governo abbia ritenuto di ampliare l'analisi, avvalendosi anche delle riflessioni e delle proposte del CNEL. Questo è il motivo per cui lo abbiamo fatto: la scelta maturata dall'Esecutivo di dare mandato a un organo di rilevanza costituzionale, terzo e specializzato, che si occupa istituzionalmente delle tematiche illustrate, è indicativa della volontà di giungere a un intervento che permetta di trovare delle soluzioni alle questioni poste in merito all'adeguatezza dei livelli salariali, con l'apporto delle parti sociali rappresentate all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ma certamente in ossequio alle disposizioni del dettato della direttiva europea

ma non obbliga gli Stati membri a istituire un salario minimo legale laddove la copertura contrattuale superi una determinata soglia, che è fissata all'80 per cento e che sappiamo in Italia essere molto al di sopra. Il tema più ampio, su cui istituzioni e parti sociali sono chiamate a confrontarsi e a individuare linee d'azione efficaci, è quello del salario dignitoso, che va oltre il salario minimo e richiede una contrattazione di qualità, capace di individuare strumenti e implementare garanzie che tutelino effettivamente lavoratori e lavoratrici. Per questi motivi, ribadisco il mio impegno affinché si seguano tutti i percorsi finalizzati a garantire livelli salariali adeguati, nel solco di un dialogo istituzionale trasparente, basato su un confronto aperto e costruttivo tra tutti gli attori coinvolti.

solo se lei avesse pronunciato tre parole semplici: salario minimo subito. Invece, mi pare abbastanza evidente, nonostante la chiarezza della sentenza della Cassazione,

Peraltro - si capiva - lei si è riferita anche al fatto che avete attribuito al CNEL un ruolo, a mio avviso, del tutto improprio e, guarda caso, proprio oggi esce la notizia che il documento del CNEL sposerebbe la linea del Governo (devo dire la verità, dal mio punto di vista è tutto

questo tentativo in atto, da parte del Governo ma non solo, di contrapporre il salario minimo alla contrattazione collettiva e al ruolo dei sindacati. Si tratta di una pessima pratica di questo Paese.

di poche migliaia di persone quando sono 4 milioni i lavoratori che guadagnano meno di 9 euro l'ora per cui francamente non mi stupisco nemmeno più di tanto. Mi dispiace che sia in atto questo vero e proprio tentativo di negare la realtà e di rendere invisibili i lavoratori poveri. Evidentemente fa parte di quello stesso furore che è stato messo in campo nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza. Fortunatamente, il 17 di ottobre, nonostante tutto, la proposta arriverà in Parlamento. Noi non ci fermiamo. Stiamo raccogliendo le firme nel Paese, continueremo a farlo e non ci arrendiamo francamente all'idea che i bassi salari debbano essere la realtà di questo Paese. Pensiamo invece che la lotta alla diseguaglianza debba proseguire e, soprattutto, auspichiamo che si applichi una volta tanto la Costituzione.

volano per lo sviluppo economico. Crede altresì che l'articolo 46 della Costituzione, che prevede nei limiti stabiliti dalla legge una partecipazione dei lavoratori

il Governo per l'attuazione piena dell'articolo 46 e della possibilità per i lavoratori di partecipare non soltanto agli utili, ma anche alla gestione delle imprese, perché pensiamo che questo sia un elemento utile a rafforzare la sicurezza nei posti di lavoro

deve affrontare nell'ottica di uno sviluppo economico e sociale che sia anche innovativo e sostenibile. Questo è quello che penso. Nel quadro normativo vigente sono previste agevolazioni sui premi di risultato in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge n. 208 del 2015 e dai successivi decreti interministeriali. In particolare, proprio la legge n. 208 del 2015, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori dipendenti, oltre alla detassazione prevede una forma di decontribuzione che si traduce in un esonero contributivo. La legge di bilancio 2023, tra le misure finalizzate a garantire maggiore potere d'acquisto ai lavoratori, prevede la parziale detassazione dei premi di risultato, con la riduzione della percentuale dal 10 al 5 per cento dell'imposizione anche sulle somme erogate e sotto forma di partecipazione agli utili di impresa. Inoltre, sempre con riferimento al coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività nelle imprese sociali, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 2017, tutte le imprese sociali devono definire, nei propri statuti o nei regolamenti aziendali, adeguati meccanismi di informazione, consultazione o partecipazione di lavoratori, utenti e *stakeholder* al fine di assicurare a questi soggetti la possibilità di esercitare un'influenza su determinate decisioni. Tra queste rientrano, in particolare, tutte quelle scelte in grado di incidere in maniera diretta sulle condizioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi forniti dalle imprese, che coinvolgono quindi più da vicino il rapporto tra le imprese e i lavoratori. Condivido l'idea di cogliere la reale opportunità, sia per i lavoratori sia per le imprese, parti della medesima comunità, di giungere a un sistema moderno di relazioni industriali. In conclusione, ringraziando i senatori interroganti per le utili e interessanti sollecitazioni, manifesto la mia disponibilità convinta, anche attraverso la costituzione di un tavolo dedicato, ad avviare una riflessione più approfondita, volta a valutare l'adozione di ulteriori iniziative legislative per valorizzare la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, magari già a partire dal prossimo disegno di legge collegato alla manovra di bilancio.

ha dimostrato sempre una capacità di ascolto, anche per le proposte che arrivano dall'opposizione, in questo caso da un grande sindacato italiano come la CISL. grazie anche per avere ricordato, indirettamente, le misure positive che ci sono nel *jobs act*. Alcuni punti che lei ha citato sono sicuramente molto importanti per i lavoratori ed hanno costituito, per noi, un elemento di importante innovazione. Dico grazie perché, purtroppo, la mistificazione politica che viene fatta del *jobs act* è molto pericolosa per il Paese. La ringrazio, inoltre, anche per aver aperto,

sia fondamentale aprire questo tavolo? Perché oggi abbiamo avuto, sul tema del salario minimo, delle risultanze. A noi non interessa quello che viene fuori dal CNEL, che per noi andava abolito, quindi non è questo il punto. Il punto è che non possiamo immaginare di intervenire sui salari delle persone aumentando le tasse al ceto medio, quindi dobbiamo dare una risposta più complessa. Il tema della partecipazione agli utili è, da un lato, capace di creare una virtuosa collaborazione tra lavoratore e impresa e, dall'altro, di sconfiggere quel pericolosissimo primato, che l'Italia ha, di un costo del lavoro altissimo, ma di buste paga purtroppo molto leggere. Ecco la complessità del lavoro dei riformisti. Un'unica notazione, signor Ministro: è trascorso un anno di lavoro dalla nascita di questo Governo. Quindi, nell'apprendere la volontà di andare verso la direzione della partecipazione agli utili di cui ella ha detto, voglio però sollecitare questo Governo a fare presto, perché il Paese non può attendere ulteriormente e questa risposta sarebbe davvero in grado di cambiare un po' le sorti dei lavoratori.

Posso dirle che non mi è parsa una buona pagina di presentazione per un'importante azienda di servizi connessa e vigilata dal Ministero del lavoro politiche sociali, perché vi si sarebbero dovute trovare le risposte, le scelte, le linee guida e i progetti, insomma ciò che caratterizza il fatto che esista una società come ANPAL Servizi SpA, che ovviamente deve rivolgersi al pubblico.

È forse in questo modo che la stessa pagina di ANPAL Servizi può continuare a produrre notizie dei progetti che erano precedentemente in atto senza dire che però c'è stato un cambiamento, la nomina di un nuovo presidente, senza che se ne abbia ragione. Vorrei ricordarle, signora Ministra, e vorrei ricordarlo a tutti noi, colleghe e colleghi, che ANPAL Servizi è un'azienda non sottoposta e non sottoponibile allo *spoil system,* quindi in realtà questo azzeramento del consiglio d'amministrazione appare esattamente come un commissariamento.

e in più abbiamo la sensazione che non sia rispettato il principio che venga diretta con un mandato legato alla disciplina e all'onore, come prevede la nostra Costituzione. Il Ministero ne è informato? Cosa intende fare?

a beneficio di tutti, che i fatti esposti nell'interrogazione e relativi a iniziative giudiziarie non coinvolgono in alcun modo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Fatta questa precisazione, rispondendo quindi ai quesiti che hanno posto i senatori interroganti, chiarisco di essere venuta a conoscenza delle notizie che riguardano l'attuale presidente di ANPAL Servizi esclusivamente da articoli di stampa e di aver poi appreso la posizione dell'interessato attraverso un comunicato stampa

per altri fatti relativi ad abuso d'ufficio e di aver dato mandato ai legali di valutare di essere immediatamente ascoltato per chiarire la sua posizione. ANPAL Servizi, come si diceva, opera nel campo delle politiche attive del lavoro ed è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale realizzando azioni e programmi in collaborazione con le Regioni e gli enti locali per migliorare le capacità di creare opportunità di occupazione, soprattutto con riferimento alle categorie deboli del mercato del lavoro. In questo senso, nell'ottica dell'importante e radicale riforma delle politiche attive del lavoro che il Governo ha intrapreso e in considerazione del ruolo che ANPAL Servizi assumerà con la riorganizzazione in atto della struttura ministeriale e il riassorbimento di ANPAL, si è proceduto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione in data 9 marzo 2023 con un decreto firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle norme È bene sottolineare che all'atto dell'assunzione dell'incarico, il presidente e i consiglieri di ANPAL Servizi non versavano in alcuna delle condizioni di inconferibilità incompatibilità rispetto all'incarico e i loro profili risultano essere rispondenti alle qualificazioni richieste, nonché alle disposizioni di legge e dunque idonei a svolgere i rispettivi mandati. Queste condizioni, allo stato attuale, non risultano essere state modificate. Il Ministero del lavoro attua attraverso le sue strutture un controllo attento e costante affinché le attività di ANPAL Servizi SpA vengano svolte sempre in osservanza della legge, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, onestà, correttezza e buona fede. Pertanto, le vicende esposte saranno seguite nel più rigoroso rispetto del lavoro della magistratura e si interverrà esclusivamente nel rispetto della legge e delle disposizioni contenute nel codice etico adottato dalla società, fermo restando il principio di garantismo che contraddistingue il nostro sistema giudiziario. Detto questo, vorrei fare mie le parole che il primo firmatario dell'interrogazione pronunciato in un intervento televisivo il 19 settembre del 2014 e che sento di sottoscrivere totalmente: il garantismo va praticato e non declamato. Mi rifaccio a queste riflessioni perché, quando si usano argomenti come quelli utilizzati nell'interrogazione, soprattutto laddove si propongono accostamenti talvolta impropri tra ipotesi di reato e in presenza di semplici avvisi di garanzia - che, è bene sottolinearlo, sono emessi a tutela dei soggetti sottoposti a indagine e non necessariamente sfociano in capi d'imputazione processuale - bisognerebbe ricordare a tutti che si è parte di uno Stato di diritto. Per il resto, sono a disposizione del Senato e anche degli onorevoli senatori e delle Commissioni per riferire sull'attività svolta da ANPAL Servizi SpA nell'ambito di tutti i tutti i processi di riforma del mercato del lavoro, che il Ministero del lavoro, a partire dal decreto-legge n. 48 del 2023, sta attuando e sta portando in avanti, non ultima la nuova piattaforma per il sistema di inclusione sociale e lavorativa su cui ANPAL Servizi sta fornendo un supporto

signor Ministro, per aver risposto a questa interrogazione, ma devo dirle che non siamo assolutamente soddisfatti della risposta, per tre ragioni che proverò a dire molto rapidamente. La prima

sono i membri del consiglio di amministrazione, che è stato decapitato da un giorno all'altro senza motivazioni: forse, anche loro avevano diritto almeno di conoscere perché, dopo pochi mesi di lavoro, non erano più nelle condizioni di svolgerlo. *(Applausi)*. Ovviamente, nel momento in cui si fanno queste operazioni, si costruisce un sospetto, che è una cosa diversa dall'essere indagati. diversa dall'essere indagati. Capisce che ci può un po' stupire - poi certamente deciderà la magistratura - il fatto che in pochi mesi di collaborazione, prima in quanto suo consulente, poi come presidente di ANPAL Servizi, il presidente sia già incappato in due grandi indagini. Capisco

delle politiche attive. Posso dirle che il Parlamento non ha partecipato e questo mi sembra un problema preoccupante, perché una piattaforma non è una riforma del mercato del lavoro.

il consuntivo dell'anno che termina ad agosto 2023, così come pubblicato dall'Istat, ci dice che per

Siamo anche al tasso minimo di disoccupazione dal 2009 (7,3 per cento). In realtà, se consideriamo gli ultimi quarantatré anni, solo tre anni hanno registrato un tasso di disoccupazione più basso di quello attuale, questo in una situazione certamente difficile, in presenza di una crescita che abbiamo la soddisfazione di constatare come sia superiore a quella media dell'Unione

per incoraggiare le assunzioni, al di là dell'aumento della produttività generale che auspichiamo prosegua in modo più abbondante nei prossimi anni per una migliorata situazione internazionale. Di fronte a questo quadro particolarmente positivo, noi del Gruppo Fratelli d'Italia le chiediamo quali ritiene siano i punti di forza che hanno permesso di ottenere tali risultati, in modo da poterli sostenere nel futuro, per l'azione del prossimo periodo

Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti. I traguardi raggiunti in materia di occupazione credo siano evidenti a tutti: come avete giustamente evidenziato, l'ultimo rapporto pubblicato da Istat ha messo in luce il *record* storico di occupazione nel nostro Paese e il fatto che il tasso di disoccupazione ad agosto 2023 sia sceso al 7,3 per cento e ci sia anche un tasso di disoccupazione giovanile in riduzione. In linea con questi dati, si segnala la crescita del numero degli occupati, che si attesta a circa 24 milioni, con un aumento rispetto all'anno precedente precedente di quasi 550.000 dipendenti e 48.000 lavoratori autonomi. Mi preme evidenziare che l'aumento dei contratti di lavoro, così importante soprattutto sul fronte di quelli a tempo indeterminato, si traduce certamente in una maggiore sicurezza economica per le famiglie italiane, che in questo modo possono progettare con maggiore serenità anche il loro futuro. Sul versante delle misure poste in essere dal Governo, il Ministero del lavoro, con il decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, ha dato attuazione alle previsioni contenute nel decreto-legge n. 48 del 2023 sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Capisco che, quando non la si riesce a cogliere, si dice che l'uva sia acerba, però basterebbe leggere il decreto di attuazione della della nuova piattaforma per il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) per comprendere dove sta la riforma e soprattutto in che modo siamo riusciti a mettere in campo azioni sinergiche per far parlare mondi che finora seguivano percorsi

e in questo primo mese di attività le domande pervenute per la misura di supporto per la formazione e il lavoro sono oltre 85.000. In questo bisogna guardare ai numeri, per dire che sono domande non solo di ex percettori di reddito di cittadinanza, ma anche di altri cittadini, cittadini, che si trovano nelle condizioni di fruire del supporto, ma non hanno un'esperienza di percezione del sussidio. Nella piattaforma abbiamo inserito, per la prima volta, una ricognizione puntuale di tutta la formazione finanziata in Italia, con una disponibilità a oggi di circa 700.000 posti nei corsi di formazione, di 100.000 progetti di utilità collettiva e di più di 70.000 proposte di lavoro, che si stanno intermediando e per le quali abbiamo già le nuove assunzioni. A questo aggiungo che, al fine di incoraggiare e sostenere l'occupazione giovanile, sempre il decreto-legge lavoro ha previsto il riconoscimento, per i datori di lavoro privati, di un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile. In relazione alle politiche attive del lavoro, il programma GOL (garanzia occupabilità lavoratori) ha raggiunto, in un anno di esercizio, un milione e mezzo di lavoratori. Su questo abbiamo anche alcune indicazioni, che ci fanno capire quali sono le qualificazioni tendenziali e le richieste in questo momento dei nuovi percorsi professionali e delle professionalità. Siamo intervenuti per ridefinire, nell'ambito del disegno di legge scuola, il percorso e il congiungimento tra la formazione professionale di natura regionale (per quanto riguarda le competenze del Ministero del lavoro) e il percorso di studi terziario oppure il mondo del lavoro. Devo dire, in conclusione, che favorire le condizioni per un mercato del lavoro più flessibile, ma allo stesso tempo sicuro, è certamente il faro della nostra azione di governo. Lavoriamo quotidianamente per favorire l'inclusione lavorativa, per rendere il mercato del lavoro più dinamico e per farlo crescere in termini di qualità. di qualità. Credo che la strada tracciata sia quella giusta. Certamente gli interventi da mettere in campo sono ancora tanti tra questi, vi è la revisione degli strumenti di politica attiva che non sono più coerenti con le necessità attuali del mondo del lavoro. Tutto questo passa però dalla lettura corretta delle dinamiche occupazionali, dalla definizione di nuove politiche coerenti - come dicevo con la transizione in atto nel mercato del lavoro e dall'esigenza di curare percorsi formativi adeguati alle richieste di nuove professionalità che vengono dal mondo delle imprese. Il tutto va unito, ovviamente, a nuove norme e strumenti che consentano un più efficace raccordo tra il mondo dell'istruzione e della formazione professionale e il lavoro, ma in questo momento ci sono a mio avviso le condizioni per far...

Signor ministro Calderone, la ringraziamo a titolo personale e a nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia. Riteniamo che le politiche che sono state perseguite, i risultati già ottenuti e quelli che ci si prefiggono

prima legge di bilancio presentata da questo Governo e di diversi altri provvedimenti. Riteniamo che sia la risposta migliore nei confronti dei cittadini italiani coloro che lavorano, di coloro che hanno cercato e trovato un lavoro nel corso di questi mesi e di coloro che ci auguriamo lo troveranno, grazie anche alle iniziative che ci ha illustrato. L'aumento della estremamente positivo, perché vuol dire che più persone hanno modo di realizzarsi attraverso il lavoro e non attraverso l'assistenzialismo, cioè in modo dignitoso, con prospettive per il futuro, facendo ciò che la Costituzione prevede, cioè contribuire al benessere della Nazione e della collettività. Questo è particolarmente significativo, dato che l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che la Repubblica si fonda sul lavoro. alle critiche e alle previsioni catastrofistiche che erano state fatte. Il lavoro - come lei ha detto, signor Ministro - è importante che sia qualificato; ci dev'essere la flessibilità per adattarsi ai tempi, ma occorre andare in una

dell'occupazione in generale crea le premesse di mercato, oltre agli interventi di altre leggi che già sono vigenti e quelle che potranno essere introdotte, per portare, per una dinamica naturale di mercato, a un aumento dell'entità infatti certamente il problema del lavoro povero, né coloro che oggi sono ancora alla ricerca di lavoro, ma il fatto di fare incontrare le esigenze delle aziende, dunque del mercato del lavoro, con la preparazione degli aspiranti lavoratori, è un aspetto estremamente importante. La ringraziamo e, a nome di tutto il Gruppo, le auguriamo buon lavoro per il proseguimento della legislatura.

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il macello di Baldichieri, azienda di 125 dipendenti situata nella provincia di Asti, ha una storia più che decennale, che a raccontarla sarebbe probabilmente troppo lunga, fatta di cambi di appalto, di subappalti e di proprietà, che in questi dieci anni si sono succedute al ritmo di una ogni due anni, quando non due contemporaneamente nello stesso anno. Parliamo di un'azienda che essendo industria alimentare ovviamente ha molto a che fare con la salute delle persone e con il tema della qualità dei prodotti. Non è un caso che tutti i processi di trasformazione alimentare abbiano regole molto più rigide e rigorose di quelle presenti in altri settori produttivi. In questi dieci anni i lavoratori e le lavoratrici di quel macello hanno avuto una grandissima pazienza, perché ogni volta si vedevano non applicati né il contratto che che spettava loro, né il riconoscimento delle loro retribuzioni e delle loro mansioni e ogni volta facevano un accordo per determinare i tempi nei quali si sarebbero applicati il contratto e le retribuzioni giusti. Il problema è che queste promesse sono state sistematicamente disattese,

quando all'ennesimo cambio di contratto, in cui veniva loro proposto per l'ennesima volta di non avere il loro contratto, né la retribuzione giusta, ma al contempo con un orario particolarmente allungato (non so se lo si sappia, ma il lavoro dei macelli non è particolarmente facile ed è sicuramente faticoso), quei lavoratori hanno detto no. Hanno detto che volevano l'applicazione del loro contratto, ciò che spetterebbe loro normalmente e il riconoscimento della loro professionalità e sono scesi in sciopero; ancora una volta, una lotta per ottenere ciò che dovrebbe essere dovuto.

Non si dovrebbe, perché la sostituzione dei lavoratori in sciopero non è permessa. È comunque assolutamente evidente la volontà, ancora una volta, di contrapporre tra di loro lavoratori in difficoltà, di ricattarli e di pensare che sia meglio che litighino tra di loro invece di dare le giuste risposte. Da qualche giorno non succede più nulla, ma noi ben sappiamo che quei lavoratori hanno avuto come risposta l'apertura della procedura dei licenziamenti collettivi. Eppure, pochi si sono sdegnati di fronte a tutto questo. Allora io credo - lo chiedo ai colleghi, alle colleghe e chiedo a lei, Presidente, di dirlo anche alla Ministra del lavoro e ai responsabili del Governo - che se vogliamo dire, come si sta dicendo in questo tempo, che la contrattazione sindacale è fondamentale e che l'applicazione dei contratti è un elemento essenziale, tanto che lo utilizzate come argomento per contrastare il salario minimo, forse la prima cosa da fare dovrebbe essere aprire un tavolo in cui ci siano quei lavoratori e quelle rappresentanze e si sancisca che il Governo interviene per far applicare i contratti nazionali di lavoro, che sono giusti e necessari. Noi lo facciamo comunque, anche se sosteniamo il salario minimo. Vorremmo lo stesso sforzo sforzo da parte di chi temo, invece, usi la contrattazione per non dare risposte ai lavoratori e alle loro condizioni.